Ciò ha permesso di snellirne l'*iter* e ci consente oggi di arrivare senza molti emendamenti e ordini del giorno a questo appuntamento.

pone al centro il superamento della crisi dell'insolvenza e non il tema del debito e della sua punizione. È una procedura che,

nella logica di ricercare fino in fondo tutte le possibilità di superare la crisi in funzione di salvare le attività imprenditoriali, i posti di lavoro e le famiglie

Garantire la continuità aziendale significa eliminare l'aspetto punitivo, che doveva esserci nella procedura concorsuale, e agevolare quindi la possibilità di recupero dell'impresa. Abbiamo sollevato solo una piccola perplessità, che forse non è nemmeno così piccola, per quanto riguarda le competenze del nuovo tribunale del fallimento, che diventerà il tribunale delle imprese.

a costo zero, ma nessun tipo di riforma della giustizia può avvenire a costo zero. Occorre un aumento degli organici o comunque una ridefinizione dei medesimi al fine di permettere la trattazione delle procedure.

a parlare il senatore Uras.

non può essere fatta senza considerare la necessità di mantenere chiarezza nelle disposizioni,

che voglio sottolineare riguarda la gestione in sede giudiziaria dei procedimenti fallimentari. L'operazione di semplificazione, con l'accentramento in un unico tribunale delle attività giudiziarie, è fortemente contestata contestata da alcune curie, in modo particolare da quelle della Sardegna. Le cito perché il presidente dell'Ordine degli avvocati ha manifestato in modo molto chiaro la contrarietà a quest'operazione di accorpamento e, conseguentemente, anche all'esclusione di agire con la competenza

anche se c'è un accenno all'ipotesi di una deroga nelle situazioni in cui, sotto il profilo logistico, non si riesce ancora a risolvere il problema di funzionamento dei tribunali. Io penso che, per quanto riguarda la Sardegna (lo dico anche al Governo), non sia pensabile passare da un regime all'altro in modo improvviso, ma che questo passaggio debba essere accompagnato da una una riorganizzazione, nonché da uno sviluppo degli organici della magistratura, perché altrimenti si rischia di intasare ancora una volta alcune linee di attività giudiziaria a danno della nostra economia, dell'interesse dei cittadini e anche dei lavoratori interessati da quelle procedure. si debba pensare anche al personale delle nostre sedi giudiziarie, che è notevolmente insufficiente. I problemi della nostra giustizia riguardano molto gli strumenti operativi in suo possesso: il personale della magistratura, gli organici dei magistrati, ma anche gli organici del personale delle sedi

che presenterò un ordine del giorno sulla questione della Sardegna, che spero sia accolto; con tale ordine del giorno si chiede che sostanzialmente il Governo pensi a gestire la fase di transizione, senza creare le disfunzioni che in altre circostanze abbiamo dovuto successivamente affrontare, perché non avevamo pensato prima a come strutturare le sedi, potenziare gli organici della magistratura, le sedi giudiziarie con personale ausiliario e tecnico professionalmente competente, compresi i livelli dirigenziali, in modo da poter consentire a quelle sedi di svolgere la propria attività, soprattutto quando tali sedi sono frutto di una riforma che incide profondamente sull'attività e sulle procedure processuali.

intervengo brevemente perché pare che ci sia un'esigenza, avvertita da tutti i Gruppi politici, di licenziare senza modificazioni questo testo che ci è pervenuto dalla Camera, sicché possa essere legge di qui a pochi giorni e contribuire a un processo di ammodernamento

fine di rendere più attuale la soluzione dei problemi relativi a condizioni di insolvenza delle medesime. Uno medesime. Uno dei miei primi impegni in Parlamento, nel 2001, atteneva proprio alla legge fallimentare. Da avvocato mi stupivo di come, nel ancora nel 2002 e nel 2003), potesse essere vigente una legge di epoca fascista, del 1942, che prevedeva, ovviamente in rapporto a quel tempo, disposizioni che andavano in direzione della tutela delle imprese. Ma i tempi erano cambiati e noi nel 2000 parlavamo ancora di di responsabilità dell'imprenditore che, in caso di fallimento, veniva visto

che, non certamente per ipotesi di condotte delittuose quali ad esempio la bancarotta fraudolenta,

diritto fallimentare. Ricordo che intervenimmo per eliminare quanto meno quel profilo sanzionatorio penale che accompagnava l'imprenditore nella procedura che lo vedeva fallito; si intervenne anche attribuendo maggiori poteri al curatore fallimentare. L'assurdo era che, con i poteri molto limitati del curatore fallimentare, "alla morte" dell'imprenditore si accompagnava la morte dell'impresa, che veniva venduta dopo anni, quando ormai le strumentazioni erano divenute obsolete e non c'era la possibilità di una riattivazione dell'impresa, sia pur con altri soggetti. Questo perché la norma prevedeva una serie di limitazioni anche nelle attività del curatore.

la decadenza. Questo va assolutamente scongiurato. Il Governo è delegato ad adottare provvedimenti

ma sostanzialmente è importante che si cominci ad allontanare dalla figura del soggetto imprenditore, titolare di un'impresa che vive una crisi economica, quella considerazione della collettività e della società

C'è un punto sul quale avrei avuto piacere di intervenire: i compensi. Ricordo una sentenza della Corte costituzionale che destò in me uno stupore straordinario.

ma ai consulenti dei giudici, a prescindere dal valore della controversia, vengono pagati i compensi attraverso le casse dell'erario. Ma la Corte costituzionale rispose in una maniera che da giovane avvocato io definii «cultura da supermercato» perché la Corte disse: qual è il problema? È prassi nei tribunali che, quando a un curatore o a un professionista si affida una curatela che non ha attivo, per cui non percepisce alcun compenso, in genere gli si affida un'altra procedura che presenta l'attivo e dalla quale può recuperare

il Governo deve fare attenzione nell'emanare i decreti relativi a questa delega, perché deve creare un esatto coordinamento con l'altro testo, che attiene alle grandi imprese in crisi. quale potrà essere la soluzione - sarà il Governo a studiarla - però, quando una grande impresa in crisi viene posta in amministrazione straordinaria,

Nel caso in cui il programma non possa essere attuato, c'è automaticamente il fallimento di ufficio dichiarato dal tribunale

altrimenti si avvia il programma di amministrazione straordinaria - che, allo stato, prevede una durata di due anni, prorogabili per altri sei mesi (quindi, due anni e sei mesi) - e, alla fine, se il programma non si realizza,

importante. Il nostro Paese sta vivendo una crisi economica molto forte e da prolungato tempo, che produce ovviamente sconquasso tra le imprese. Il tema del diritto fallimentare o, in questo caso, delle crisi e delle situazioni di insolvenza è enorme: si va, purtroppo, dalla piccola circostanza di paese, dove l'artigiano si trova di fronte a una situazione insormontabile, fino ad arrivare alle grandi crisi industriali, come quelle che stiamo vivendo e vedendo in questi giorni con l'ILVA o altrove. Si tratta di realtà estremamente differenti ed è anche difficile accostarle.

dalle situazioni nelle quali gente onesta si trovi disgraziatamente a vivere condizioni di insolvenza e di incapacità ad affrontare i debiti che un mercato instabile instabile rende pesanti come macigni. L'obiettivo deve essere rivolto a questi ultimi soggetti che operano nel mercato e che, rischiando in proprio, si trovano nell'incapacità di assolvere agli impegni presi. Queste crisi devono essere risolte senza che vi sia

dati da chi in quella casa dovrà andarci ad abitare: quando questi soggetti vanno incontro a situazioni di insolvenza o di difficoltà, a quel punto è una catastrofe non solo per loro, ma anche per tutti coloro che vi sono collegati. Chi perde la casa su cui ha investito tutti i risparmi non riesce più a trovare una soluzione per uscirne. Si tratta di situazioni veramente complicate.

Se il Governo attuerà la delega velocemente o se lascerà passare il tempo, scavalcando la prossima legislatura, può fare la differenza.

Non si può attendere ulteriormente nel dare soluzioni alternative rispetto a quello che oggi brutalmente si chiama fallimento. Abbiamo un sistema normativo farraginoso, composto da sovrapposizioni e stratificazioni che nel tempo hanno reso tutto più frammentario; anziché rendere le soluzioni più facili, le hanno rese più complicate.

Vedo che sopra il testo - giova ricordarlo - vi sono le firme del ministro Orlando e, ancora, del ministro Guidi. Governo, di tempo ne è passato parecchio! Su questi provvedimenti bisogna essere molto più veloci. Ci sono delle criticità, che sono state sollevate dagli avvocati e ovviamente dalle parti sociali. Siamo convinti che non sia ancora il provvedimento ideale, ma siamo certi che questo possa essere un provvedimento utile, se nelle deleghe il Governo terrà conto di tutte le considerazioni emerse dagli ordini degli avvocati, dai civilisti, dai penalisti, dai professionisti, da tutti coloro che sono interessati e che sappiamo hanno indirizzato al Governo le proprie riflessioni.

si occupa di crisi di impresa, una disciplina estremamente delicata, perché riguarda il funzionamento del tessuto economico del nostro Paese, nei momenti in cui proprio quel tessuto si trova in difficoltà. I tempi appena passati e la crisi che ha colpito l'Italia - e non solo - hanno dimostrato la necessità di adeguare la normativa, sia sostanziale che processuale, allo scopo di affrontare al meglio le difficoltà dell'impresa, preservando, per quanto possibile, la capacità produttiva del sistema. L'obiettivo del disegno di legge al nostro esame, l'Atto Senato 2681, è dunque quello di intervenire in modo organico su una disciplina che risale, nei suoi capisaldi, alla legge del 1942,

Siamo in un'epoca in cui la rapidità, la velocità e la dinamicità dei fenomeni economici sono tali che spesso il legislatore è incapace di tenerne il passo: tentare di rispondere a tale dinamismo con una disciplina puntuale rischia di essere fatica inutile e priva di effetti, se non dannosa per quella ricchezza che si vorrebbe preservare. allora giungere - ed è questo l'obiettivo della riforma - a discipline organiche, entro le quali sia possibile individuare principi chiari, che possano offrire agli interpreti, anche di fronte a fenomeni nuovi, la possibilità di ricavare la norma da applicare al caso concreto, in modo che non sia necessario rincorrere in continuazione i fenomeni economici, ma sia possibile, l'appunto, da principi chiari, entro leggi omogenee e con una propria coerenza interna, ricavare quelle regole che consentano agli interpreti di intervenire, anche a fronte delle modifiche repentine della società e dell'economia. Questo è, quindi, il grande obiettivo che va assegnato alla riforma organica della disciplina della crisi di impresa, parte nevralgica e delicata del nostro sistema giuridico, proprio perché interessa il sistema economico, nel momento in cui affronta le situazioni di difficoltà.

delle loro ragioni di credito e in tempi più veloci possibili. È inoltre presente l'interesse della società, dell'impresa in stato di crisi, che riguarda l'impresa in sé, ma anche il tessuto economico complessivo generale, che è interessato a non disperdere i valori rappresentati da quell'impresa, primo fra tutti quello occupazionale. È anche presente l'interesse delle imprese sane ad evitare che il prolungarsi della crisi di imprese in stato di decozione,

infatti, lasciamo sul mercato troppo a lungo imprese che, invece, sono in condizione di pre-insolvenza o, comunque, di crisi conclamata, rischiamo di alterare anche il meccanismo di funzionamento del mercato. La legge fallimentare, come è stato detto, negli ultimi dieci anni ha subito diversi rimaneggiamenti, ma i ripetuti interventi normativi, motivati il più delle volte dal dissesto di singole imprese e quindi da necessità occasionali, erano non sempre connotati dal requisito dell'urgenza, per cui è diventato sempre più necessario intervenire con una disciplina che portasse una razionalizzazione del sistema delle procedure. Il provvedimento di cui oggi discutiamo è innovativo sotto diversi profili e ruota attorno ad alcuni principi cardine che sono riassumibili nei seguenti punti: la centralità del fenomeno dell'insolvenza anche nella sua accezione di crisi rispetto alla qualificazione soggettiva del debitore, consentendo in tal modo a tutti i debitori di poter accedere agli istituti finalizzati alla sistemazione dei debiti; gestione della crisi e dell'insolvenza del gruppo; prevenzione dell'insolvenza sin dai primi segnali di crisi nell'ottica della conservazione dei valori aziendali; responsabilizzazione degli organi di *governance* e dell'imprenditore; residualità della liquidazione, intesa come ultimo strumento per comporre la crisi; sostituzione del termine «fallimento» con quello di «insolvenza». Con questo provvedimento sono state introdotte soluzioni che, fino ad oggi, erano sconosciute nel nostro ordinamento. Una delle novità più rilevanti della riforma è l'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che assolvono all'importante funzione di far emergere in maniera tempestiva lo stato di crisi di chi non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. Nell'ottica di incentivare l'emersione anticipata dalla crisi e, dunque, il momento in cui si riscontra la probabilità di futura insolvenza, l'articolo 4 delega il Governo ad introdurre le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Questa procedura rappresenta un momento di rafforzamento delle possibilità di successo di un programmato e strutturato percorso di risanamento; un percorso che l'impresa, specie se di piccole dimensioni, in tempi che non devono essere lunghissimi, dovrebbe intraprendere facendosi affiancare da soggetti professionisti del settore con esperienza e provata professionalità. Non solo, ma è fondamentale che, in questo quadro, anche la magistratura sia in grado di espletare in maniera esaustiva il proprio ruolo, data anche la natura chiaramente specialistica delle competenze giuridiche in ambito di procedure concorsuali. Si prevede, inoltre, il coinvolgimento di molti enti pubblici, come gli enti di riscossione e di previdenza che diventano parte attiva nel monitorare in modo costruttivo l'andamento economico-finanziario dell'imprenditore. È fondamentale che siano portati alla luce tempestivamente comportamenti che, a lungo andare, si rivelerebbero estremamente dannosi per l'azienda, anche per impedire che - con il tempo - l'impossibilità di far fronte, da parte dell'azienda, alle proprie obbligazioni, abbia un effetto domino su tutti gli altri soggetti con i quali quali essa opera, a cominciare dai creditori e proseguendo naturalmente con i lavoratori e con tutte quelle imprese che fanno da satellite alle imprese in crisi. Ma l'innovazione non si ferma alla fase preventiva di allerta, finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e alla sua risoluzione assistita, come ricordava poc'anzi anche il senatore Falanga. Anche il vocabolario cambia, perché nessuno potrà essere più apostrofato come «fallito» e scomparirà anche la parola «fallimento» e la relativa procedura, che verrà sostituita dal termine «liquidazione giudiziale». Si semplificano le regole processuali, prevedendo l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; si individua il tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando le procedure di maggiori dimensioni al tribunale delle imprese (sezione specializzata a livello del distretto di corte d'appello). Consentitemi un commento, per così dire, lo sforzo di specializzazione, cioè di risposta competente e veloce al problema, deve essere compiuto proprio da tutto il mondo della giustizia e della giurisdizione. Lo sforzo è stato chiesto all'avvocatura, ma uguale necessità deve essere anche a carico della magistratura; e spesso tale sforzo non viene fatto. si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella della liquidazione giudiziale. Cambia dunque anche la procedura, con l'eliminazione di quella fallimentare e con il curatore che diventa il "*dominus*" di quella nuova con poteri rafforzati e il possibile sbocco di un concordato di natura liquidatoria. In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione. Dovrà, inoltre, essere data priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come ultima *ratio*. Rivisitata anche la disciplina dei privilegi, ritenuta ormai obsoleta, e previsto un sistema di garanzie mobiliari non possessorie. Nella delega si facilita l'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione del debito; si rivisita, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo, considerato ad oggi lo strumento più funzionale tra quelli vigenti; si elimina come procedura concorsuale la liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; si prevede una esdebitazione di diritto per le insolvenze di minori dimensioni; si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento; colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare, si introduce, infine, una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese. Concludo, auspicando che, grazie al lavoro comune di Governo e Parlamento, e ringrazio qui ancora una volta i colleghi senatori che hanno privilegiato la rapida approvazione alla propria legittima aspirazione

che gravitano intorno ad un'impresa validi strumenti per superare il momento di difficoltà e continuare ad essere protagonisti nel mondo imprenditoriale e volano per l'economia del nostro Paese.

anche in questo caso ci avete un po' messo lo zampino, perché, su uno stile derivante da un approccio molto globalizzato, che è molto vicino a quello del vostro ministro Calenda, abbiamo usato un po' un metodo cinese. quasi tutti sappiamo, infatti, che nella lingua cinese la parola crisi non esiste, quindi l'ideogramma che i nostri amici cinesi usano per identificare la crisi in realtà, significa nuove opportunità. Quindi, secondo lei noi stiamo facendo questo. stiamo facendo questo. Però, alla base delle amministrazioni straordinarie, dei concordati fallimentari, delle liquidazioni, ci sono delle persone e ci sono delle famiglie. E io non credo che a queste famiglie e a queste persone basti semplicemente cambiare il nome a quello che sta avvenendo per poter portare un'onda di ottimismo. E perché dico questo? Lo dico perché il Ministero dello sviluppo economico,

Un punto fondamentale, che ormai non attiene più al provvedimento, è il fatto che è stata sottratta al controllo parlamentare

Guarda caso, proprio in questo provvedimento si inserisce una norma, quella che poi è stata varata con decreto ministeriale dal ministro Calenda, per nominare una commissione di esperti che scelga i suoi commissari. Tra i tre esperti c'è il già citato Enrico Bondi. In questo alveo si inserisce il tema dei concordati fallimentari e dei compensi d'oro dei commissari

su tutti un caso importante che è stato gestito dal Ministero, motivo per il quale era inserita nel provvedimento la norma per la riappropriazione da parte del Parlamento della gestione di determinate crisi.

specializzata nel diritto fallimentare (stiamo parlando di circa otto magistrati e sono pochi i tribunali che possono permettersi una specializzazione di questo tipo), significa

L'accorpamento potrebbe sembrare apparentemente uno snellimento e una ottimizzazione, ma tutto questo va scapito del cittadino e delle imprese che dovranno rivolgersi a sezioni specializzate che molto probabilmente

nell'alveo di quella riforma della geografia giudiziaria che è iniziata con la chiusura di un numero elevato di tribunali e che ha colpito tutti i nostri territori. Chiunque di noi, infatti, è stato intercettato da questo da questo problema, perché ognuno di noi ha un suo territorio che vuole ovviamente, giustamente e legittimamente tutelare.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge delega che oggi andremo ad approvare rappresenta, pur con qualche aspetto ancora migliorabile, una novità positiva. Innanzitutto perché tiene conto che la crisi economica che ha attanagliato il nostro Paese per molti anni ha provocato molte situazioni di crisi aziendali che, non sempre colpevolmente, hanno portato alla richiesta di adesione al concordato preventivo, alle dichiarazioni di liquidazione coatta o di vero e proprio fallimento. Per questo giudichiamo positiva la volontà del provvedimento di promuovere ogni iniziativa che porti l'azienda ad evitare il fallimento. A partire dalla sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale", alla sostituzione della dichiarazione di fallimento d'ufficio con i concetti

Bene quindi tutte le misure che incentivino gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, così come accogliamo positivamente i principi e i criteri fissati per la riforma del concordato preventivo e la disciplina dei compensi dei professionisti incaricati delle procedure. Tra le deleghe affidate al Governo con questo provvedimento vi è anche la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e il sistema dei privilegi e delle garanzie. Un ambito strettamente connesso con il cosiddetto concordato preventivo, che adesso diventa solo concordato in continuità, materia sulla quale io, ed altri colleghi, siamo intervenuti in passato con diverse iniziative per chiedere una revisione dello strumento, ed evitare i suoi abusi o un utilizzo distorto, a danno dei creditori. Mi riferisco in particolare al cosiddetto concordato in bianco, utilizzato troppo spesso come *escamotage* per dilazionare nel tempo i pagamenti ai creditori, se non addirittura per eluderli, attraverso la costituzione di *new company* che rilevavano l'attività. I dati che abbiamo la dicono lunga su come molti operatori hanno utilizzato il concordato a cui hanno avuto accesso in maniera indiscriminata e senza filtro alcuno, aziende che da un lato volevano solo dilazionare o eludere i pagamenti, altre che invece erano già decotte e non risanabili in alcun modo. È giusto quindi intervenire per rivisitare a fondo uno strumento che, per quanto nato con le più nobili intenzioni, ha prodotto situazioni sconcertanti. Sconcertanti perché, attraverso il concordato, in molti casi, il più furbo o il più incapace si è rifatto o ha scaricato le sue difficoltà sulla pelle dell'onesto. L'azienda che era in crisi, in alcuni casi semplicemente per una sua cattiva e dissennata gestione, si è rifatta sull'azienda che produceva, che lavorava, che sapeva gestirsi in maniera accorta e responsabile. Come autonomisti siamo intervenuti molte volte sull'argomento sia attraverso ordini del giorno che con emendamenti approvati nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare. Da ultimo ho presentato il disegno di legge n. 2211,

In definitiva, dobbiamo rendere il concordato in continuità uno strumento equilibrato tra diritti dei creditori e necessità di non disperdere importanti patrimoni aziendali, perché quello che è accaduto in questi anni è qualcosa di inaccettabile.

perché anche oggi sono purtroppo in atto speculazioni micidiali con creditori che non vengono pagati e aziende che rilevano le ditte in difficoltà, che producono utili notevoli. Credo allora che anche i diritti dei creditori prima del concordato debbano essere

La prima di esse è emersa in alcuni interventi, ma vorrei fosse molto chiara, al netto di alcune osservazioni che sono arrivate dal dibattito e che hanno teso a banalizzare il concetto. esame è impostata su un criterio assolutamente rivoluzionario rispetto al quadro precedente. La crisi d'impresa non è assunta sotto il profilo della penalizzazione dell'imprenditore, le cui responsabilità verranno accertate. L'obiettivo che si pone la nuova legge fallimentare è quello di cercare di verificare tutte le possibilità per superare la crisi, per evitare che il Paese perda un'unità imprenditoriale e che si perdano posti di lavoro. Credo che questo sia assolutamente decisivo penso che chi ha frequentato i tribunali sappia cosa vuol dire questo rispetto all'attuale procedura fallimentare. Con quest'ultima il debitore diventa diventa un «appestato», non ha più il diritto di parola e deve subire tutte le conseguenze di una procedura che mira ad che mira ad accertare le responsabilità e non si occupa, se non in misura secondaria, dell'impresa e del suo destino. Nella logica di questo provvedimento, invece, partendo dallo stato di crisi, si cerca di verificare le condizioni per salvare l'impresa e quindi, in prospettiva, le *chance* che l'imprenditore andato in crisi deve avere nella sua vita futura, senza rimanere penalizzato da una vicenda

della situazione da parte sua. Credo che l'esempio sia estremamente attuale, nel senso che stiamo uscendo da una crisi decennale che, in alcuni settori, ha determinato

lo stesso Sottosegretario - si avrà grande attenzione a bilanciare adeguatamente le responsabilità proprio in questa prospettiva. C'è un secondo tema che è stato

delle imprese dello stesso gruppo e una trattazione congiunta del loro fallimento può consentire di evidenziare gli intrecci, le operazioni illecite e le responsabilità trasversali all'interno del gruppo di imprese.

in Aula questa riforma e procedere alla sua approvazione. Anche dagli interventi svolti questa mattina nel corso della discussione generale emerge una sostanziale condivisione dell'approccio culturale che caratterizza questa riforma che - ricordiamoci - interviene su un regio decreto del 1942 e consente il superamento dello stigma del fallimento,

un equilibrato contemperamento tra le esigenze di specializzazione e quelle di prossimità e adeguata rispondenza nei tempi della nuova strutturazione territoriale,

perché l'approvazione della riforma oggi consente al Governo di esercitare la delega in tempi compatibili con la fine della legislatura.

che riguarda il dispositivo. Nel primo capoverso del dispositivo si chiede di sostituire le parole «consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori» con «introducano nell'ordinamento misure di tipo premiale in relazione alla responsabilità degli amministratori». Si chiede inoltre di sopprimere il secondo punto del dispositivo.

sostituire le parole «includendo quelli con il circondario di almeno 200.000 abitanti» con le parole «e, salvo circostanziate e specifiche ragioni, con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti».

e analisi dei dati disponibili; impegna il Governo: a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, in via tendenziale, in numero non inferiore a due per ciascun distretto di Corte di appello, al fine di impedire che la riforma comporti un rallentamento dei tempi delle procedure conseguente ad un esponenziale e non proporzionato incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di grandi dimensioni,

avremo un Parlamento che dà due o tre interpretazioni diverse alla stessa questione.

il criterio del «non inferiore a 200.000 abitanti»; dall'altro, il criterio minimo dei due tribunali per ogni Corte d'appello. Io sinceramente eviterei di cancellare uno dei due criteri, perché non sono tra loro in contrasto e incompatibili.

Signora Presidente, se il senatore Caliendo è d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno

unanimemente condivisa l'esigenza di non concentrare solo sui grandi tribunali, poiché sarebbe un rallentamento. Questa mi sembra una razionalizzazione positiva.

anche il sottoscritto e gli altri colleghi del Gruppo sono tentati, come ha fatto il collega Lucidi, di chiedere di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno G2.101 (testo

la situazione, che evidentemente è uno dei punti cruciali visto che c'è un interesse diffuso alla questione della geografia giudiziaria dei nuovi tribunali

Casson e Caliendo, prende questo impegno - per quanto possa valere un ordine del giorno - di trovare soluzioni alternative prendendo in considerazione la popolazione residente nel circondario o il numero di tribunali per corte d'appello, forse sarebbe il caso di riconsiderare il tutto adesso e mantenere le competenze territoriali come sono attualmente, prevedendo misure ragionevoli di adeguamento del personale. Non chiedo, pertanto, di aggiungere la mia firma agli ordini del giorno che stanno raccogliendo tanto consenso, seppur condivisibili per alcune parti,

che hanno concentrati in poco spazio milioni di abitanti - come, ad esempio, Roma

in grande difficoltà da questo punto di vista. L'ottica che aveva prima lo Stato - lo Stato costituzionale - era quella di avvicinare il servizio al cittadino,

tuttavia rilevare che tra i due ordini del giorno c'è una differenza così sostanziale che non rende possibile un'ipotesi di tal genere. Il senatore Casson propone di implementare l'organico dei giudici delle sezioni fallimentari già attualmente esistenti con la partecipazione, all'interno, di figure professionali quali avvocati che abbiano maturato una certa esperienza e dottori commercialisti che avessero

fallimentari; tra l'altro, al di là della competenza tecnica, una procedura fallimentare, come noi sappiamo, è ricca di eccezioni, che sono di natura squisitamente processuale e che esigono una competenza specifica, non già soltanto in materia commerciale, ma anche in materia di diritto processuale civile.

Probabilmente manca l'esperienza sul territorio negli uffici giudiziari; ci sono poi piccoli tribunali che non hanno un organico tale da poter garantire l'istituzione di una sezione specializzata in materia fallimentare. Prevedere, invece, come fa il senatore Caliendo, di sollecitare il Governo a individuare quei tribunali che possano garantire una elevata professionalità e un'adeguata istituzione delle sezioni fallimentari mi sembra la via più ragionevole. Pertanto, con tutto il Gruppo

che l'ordine del giorno a firma Caliendo è di facile attuazione e va nella direzione più ragionevole e più celere, che il

non avevo la possibilità di ricevere appoggi sul mio ordine del giorno e ho tenuto conto della possibilità che si affermasse un principio di allargamento, quanto più è possibile, delle sezioni per l'impresa, perché altrimenti ci si riduce in un vicolo troppo stretto. [**Presidenza del vice

sia contrario su tutti gli emendamenti.

mira ad introdurre specifiche conseguenze premiali o sanzionatorie a seconda del comportamento dell'imprenditore. L'importante è che sia chiaro che non parliamo di due distinte procedure, ma solo di conseguenze

G2.102 il parere rimane contrario, perché nega il criterio della specializzazione del giudice, che è un criterio peraltro richiesto anche in sede europea.

chiede di lasciare invariati gli attuali criteri di distribuzione territoriale delle sedi. Il Governo chiede al senatore Uras di condividere invece gli ordini del giorno G2.101 (testo 3) e G2.103 (testo 2), che vanno incontro alla stessa esigenza e cercano di contemperarla con l'esigenza di specializzazione, che è quella contenuta nella delega.

se noi trattiamo l'Italia come se fosse una cosa unica e non riusciamo a capire che c'è una diversità territoriale, che c'è una diversa condizione rispetto ai processi di spopolamento, che c'è una diversa condizione rispetto all'organizzazione dei servizi generali, noi non rispettiamo il senso dell'articolo 5 della Costituzione, che impone allo Stato di operare il decentramento dei servizi pubblici per garantire l'uguaglianza tra i cittadini del nostro Paese.

ad assicurare, in conformità agli strumenti offerti dalla disciplina vigente, il monitoraggio della fase preventiva anche delle società quotate in mercati regolamentati e delle imprese definite grandi dalla normativa UE».

per le nomine, da parte dei professionisti, delle varie curatele o delle procedure disciplinate dall'articolo 7. È un emendamento che vuole incidere su quelle realtà, così frequenti

di incancrenimento di equilibri di nomina all'interno dei singoli fori, che sarebbe opportuno scoraggiare con criteri ben più chiari che impongano una rotazione nell'affidamento degli incarichi. L'emendamento, nella sua lettera *a-ter),* prevede anche che sia pubblicato un elenco su Internet e che i professionisti nominati siano sottoposti a valutazione da parte del tribunale in modo da poter garantire anche la qualità

di un impegno «a valutare l'opportunità di considerare eventualmente».

Signor Presidente, come già rilevato in sede di discussione generale, il disegno di legge

Ricordiamo che le procedure concorsuali nascevano in origine con l'unico obiettivo di assicurare la cosiddetta *par condicio creditorum*. Il fallimento interveniva proprio al fine di permettere che tutti i creditori potessero essere trattati in egual maniera e poter così soddisfarsi sui beni dell'azienda fallita.

se desta perplessità il fatto che questo tipo di intervento debba avvenire a costo zero. Infatti, come previsto nell'ultimo articolo del disegno di legge, parrebbe che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si comprende allora come questi organismi

di applicazione e di emanazione dei decreti legislativi mai si sa quale possa essere la sorte. Le leggi delega hanno nascosto tante insidie e anche qui ci troviamo

C'è un problema che riguarda la competenza di quello che vorrebbe essere il nuovo tribunale dei fallimenti, quasi tutto concentrato presso le sedi dei tribunali delle imprese.

era sorto il problema di come riuscire a contemperare i due diversi interessi: da una parte, avere una magistratura specializzata in diritto fallimentare e suggerire quindi suggerire quindi un percorso di concentrazione del tribunale; dall'altra, assicurare quel contatto che c'è sempre stato fra l'avvocatura, i cittadini e il tribunale dei fallimenti, così come dislocato nelle varie sedi provinciali,

dati, che per certi versi possono anche inquietare. Attualmente le sezioni specializzate hanno un carico di lavoro che sta aumentando

tra l'altro, è molto costoso, visto che il contributo unificato per radicare una causa è il doppio rispetto a una domanda di pari valore in un tribunale ordinario), i tempi della definizione purtroppo hanno subìto rallentamenti. Se nel 2014 il 74 per cento delle cause era concluso in un anno, nel 2016 - cioè solo due anni dopo - si è già calati al 57 È questa, la problematica. Non andiamo forse a caricare il tribunale e ad appesantirlo di procedimenti che andranno a vertere quasi esclusivamente sul tribunale? Ma soprattutto, come tra l'altro è stato evidenziato negli ordini del giorno, dividere le varie competenze, come si vuol fare nel disegno di legge, fra il tribunale dei fallimenti, che andrà quindi nei capoluoghi di Regione oppure nei tribunali più importanti, per quelle che restano, il tribunale ordinario, non potrà creare problemi applicativi o più problemi rispetto a quelli che si vogliono risolvere? In buona sostanza, ci troviamo di fronte a queste consuete, continue problematiche che riguardano la distribuzione dei carichi. Lo abbiamo visto anche in sede di riorganizzazione della geografia giudiziaria: per cercare di snellire, si è appesantito; per cercare di risolvere, si sono creati ulteriori problemi. Poi, alla fine, in Italia si accetta tutto e si fa passare un po' tutto,

presso il tribunale delle imprese, futuro tribunale quindi anche dei fallimenti; se tutti siamo stati d'accordo e se tutti li abbiamo votati, significa che la legge ha un problema. Quindi significa che si sarebbe dovuta modificare la legge su quel punto, altrimenti non si vede perché ci sia un accordo globale sugli intenti

problemi ci potranno essere. Occorre una vicinanza, come abbiamo sempre detto. Oggi parliamo di autonomia, come stiamo facendo noi in Lombardia e in Veneto per il *referendum*,

mettere chilometri di distanza significa non solo aggravare i costi, ma anche creare una distanza di verifica e controllo.

dico subito che, trattandosi di una legge delega, il giudizio si dà sul contenuto della delega e sui principi, perché, come qualcuno ha detto poco fa,

ben settantacinque anni fa, in una direzione di cui si sentiva veramente bisogno sul territorio e in tutti i tribunali italiani. Si tratta di una modifica di non poco conto, non solo per l'ampiezza della modifica, ma anche per l'approccio culturale e di politica giudiziaria.

quanto era difficile dire ad una persona che era fallita, magari non alle tante persone che con quel fallimento poi concretizzavano ipotesi di bancarotta fraudolenta o quant'altro, ma alle persone che avevano avuto realmente delle difficoltà, spesso a gestire imprese individuali, quindi senza alcuno schermo e senza alcuno scudo.

è proprio l'ottica: non si tratta più di penalizzare l'imprenditore che non ce la fa, ma di mantenere le conseguenze del caso (anche le più gravi, nel caso di imprenditori disonesti) e al contempo di tutelare le aziende

modifica quindi non è lessicale, né quando si parte dal fallimento per arrivare alla liquidazione giudiziale, né quando si parte dallo stato di dallo stato di insolvenza per arrivare invece alla definizione dello stato di crisi, che ovviamente viene prima dello stato di eventuale futura insolvenza.

tra un debitore e un altro, con casistiche su cui la giurisprudenza ha dovuto fare strada e aiutare i tribunali fallimentari a fallimentari a capire chi avevano davanti, quanto di poter assoggettare alla procedura di accertamento dello stato di crisi, e quindi di insolvenza, ogni categoria di debitore. Anche questo è un punto di qualità. Segnalerò soltanto i punti che mi sembrano di particolare qualità

ma io non sarei troppo rigida in tutto questo, perché l'affidamento degli incarichi è attribuito a un tribunale e nei tribunali di frontiera, rispetto a fallimenti difficili e complessi, rispetto a fallimenti di imprese gestite al di fuori della legalità o da soggetti che, magari con lo scudo della legalità, gestiscono imprese finanziate con soldi riciclati, spesso è difficile anche trovare dei curatori. Quindi ben venga l'albo, perché questo eviterà che sul territorio si faccia incetta di fallimenti ed eviterà tante storture che abbiamo visto sul territorio. Ben vengano anche i criteri, ma con una certa elasticità mentale, perché sappiamo che si tratta di patologie delle imprese, si tratta di stati di crisi e di insolvenza, si tratta di imprese che non vanno bene. Sappiamo anche - e lo sa bene la legge delega, quando precisa che rimangono inalterati i reati fallimentari - che nella maggior parte dei casi, quelli che più hanno affaticato non solo i tribunali, ma anche

circoscritto i poteri e i doveri di questo tipo di professionisti. Secondo me le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, di cui all'articolo 12, dà risposte importanti. Infatti, molto spesso, negli stadi fallimentari, abbiamo assistito a gente che di fatto è fallita in proprio ed ha perso ogni patrimonio, perché aveva investito i propri risparmi in appartamenti che non sono mai stati costruiti. Complessivamente il nostro giudizio è positivo. Manca qualche norma, che d'altra parte non rientrava nella legge fallimentare, bensì nella legge n. 95 del 1979, ma voteremo favorevolmente.

Signor Presidente, accettando l'invito ad essere sintetico, esprimo il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie, Partito Socialista Italiano e MAIE, consapevole di portare a termine un provvedimento importante. Noi esprimiamo un giudizio molto positivo: si tratta di una buona legge, attesa da anni, che cambia completamente l'impostazione normativa passando da una fase sanzionatoria nei confronti delle imprese in difficoltà e da un atteggiamento negativo a un completo ribaltamento dell'impostazione, avendo come punto di riferimento principale il mantenimento in vita dell'impresa, in quanto non soltanto patrimonio dei possessori degli imprenditori, ma anche patrimonio e ricchezza del Paese. C'è da considerare tra le misure importanti previste, anche se penalizzante nei confronti delle piccole imprese, l'introduzione dell'obbligo del revisore dei conti anche per le imprese minori, quelle che hanno più di dieci dipendenti e più di 2 milioni di fatturato annuo, l'adozione del criterio dell'azione preventiva, in modo tale da evitare le crisi e portare anche le piccole imprese, che spesso sono carenti da questo punto di vista, a una gestione efficiente e razionale, in linea con i princìpi di buon governo dell'impresa. Certamente, rimane il punto critico della scelta dei curatori e degli amministratori giudiziari perché sicuramente manca la valutazione di un criterio di equità di peso degli incarichi e, in questo senso, si auspica che il Governo, attraverso la delega, eserciti una puntuale regolamentazione della materia onde evitare azioni non conformi al principio fondamentale della terzietà dell'azione del giudice rispetto agli incarichi, in modo tale da evitare favoritismi che anche le cronache hanno messo in risalto. La situazione penale, dal punto di vista della responsabilità degli amministratori, rimane invariata. Si tratta, complessivamente, di un buon provvedimento, al di là delle critiche che sono state mosse, più spinte da una posizione pregiudiziale che da una questione di merito. Credo che il Paese avesse bisogno da tempo di questa legge e oggi noi, approvando il testo che ci è arrivato dalla Camera, concludiamo un *iter* di cui tutti dobbiamo essere onorati, perché dotiamo il nostro ordinamento, pur nelle difficoltà di questa legislatura, di un provvedimento sicuramente indispensabile per rendere il nostro Paese moderno anche da questo punto di vista.

commento sui tratti salienti del disegno di legge che stiamo approvando. Il primo argomento di positività è uno scenario

dettati in diverse circostanze, soprattutto dalle emergenze, e non avevano una complessiva razionalità e organicità. A questo si pone rimedio con la disposizione di legge che stiamo approvando. La *ratio* è stata ampiamente dibattuta, ma mi fa piacere poterla rimarcare: la possibilità, pur in presenza di crisi aziendale, di proseguire l'attività dell'azienda, superando la crisi, con una serie di interventi che partono dalla procedura di allerta per affrontare la crisi medesima con l'istituzione di una procedura una procedura particolarmente interessante e utile e, cioè, la composizione assistita per favorire il superamento dell'insolvenza. Il fallimento è sostituto dalla gestione della crisi d'insolvenza. La legge fallimentare risale al 1942, novellata poi nel 2006 e modificata diverse volte, ben sette da allora. Il quadro, quindi, è composito.

dall'Europa e dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale. È istituito, come rimarcato da altri colleghi e mi preme sottolinearlo, il concordato di gruppo, gruppo, argomento di grande rilievo per evitare casi distorsivi, già verificatisi, di aziende che facevano fallire una componente dell'insieme, in danno ai creditori, conservando completamente l'utilità dell'operazione, senza subirne le conseguenze. La composizione assistita è forse la vera novità di questo intervento. Prevede un monitoraggio preventivo, in modo da contenere i danni e salvare l'azienda. Il concordato preventivo è oggetto di attenzione; è stato finalmente espunto dalla legislazione il concordato liquidatorio puro, puro, ammesso solo quando il debitore proponente apporta anche altre risorse esterne, oltre a quelle esistenti, con un apprezzabile incremento del patrimonio, che consenta comunque il soddisfacimento di almeno il 20 per cento della massa creditoria inevasa.

prevedendo il concordato misto, con una connessione tra la continuità aziendale e una contemporanea liquidazione parziale delle insolvenze. È stata riservata una particolare attenzione ai poteri del curatore, che è il vero *dominus* della liquidazione giudiziaria, con precise norme che ne rinforzano e ne chiariscono il ruolo. È previsto anche il diritto di informazione del debitore, che nella legislazione vigente era, invece, ignaro di quanto accadeva al suo patrimonio, consentendogli quindi di rimanere in contatto con la realtà che ha creato, ancorché vulnerata da crisi aziendale, nell'ipotesi che possa La materia della composizione della crisi e dell'indebitamento risale alla legge n. 3 del 2012 e ha avuto, in termini di esperienza, risultati piuttosto lacunosi.

che ha portato, negli ultimi dieci anni, a una stratificazione normativa, quindi a una difficoltà da parte di chi deve gestire l'intero impianto e a una difficoltà per i creditori chirografari ad essere soddisfatti. poi l'inserimento, all'articolo 11-*bis* (è un dettaglio significativo), del controllo di legalità da parte del notaio, notaio, soprattutto per rimediare alla disapplicazione della garanzia fideiussoria a favore dei promittenti acquirenti dell'immobile, che non era sostanzialmente applicata.

organi di controllo nel caso in cui vi sia un'incongruità di rapporto tra il patrimonio della società e l'indebitamento. Infine, l'ultimo aspetto, quello forse più innovativo e più importante, anche *de iure* *condendo*: l'istituzione di un giudice specializzato, che possa seguire, per competenza, esperienza, funzionalità, capacità di intervento, con più appropriata professionalità i casi di questo genere. Occorre segnalare al Governo che l'Assemblea si è espressa ampiamente a favore in questa direzione. Il tribunale delle imprese ha funzionato ed è una delle riforme più significative che abbiamo introdotto durante questa legislatura. È proprio in questo scenario e in questo contesto che devono essere individuate le risorse organizzative, professionali, gestionali del sistema giustizia per l'affidamento al giudice specializzato della gestione dei casi di insolvenza, affinché possa utilmente essere applicata questa norma che, ripeto, come dicevo all'inizio, ha il nostro pieno accordo e il nostro voto favorevole. *(Applausi del

che il Governo le ponga in essere e che il Parlamento, come naturale, controlli. Anche la delega, se usata in maniera corretta e non abusata, è infatti uno strumento indispensabile della democrazia. Venendo al merito, c'è nel provvedimento uno sforzo semantico, per cui il fallimento ora si chiama liquidazione giudiziale. Potrei fare dell'ironia su questo riformismo semantico, ispirato da un politicamente corretto buonista,

che, in questo caso, si sia voluto scindere il termine fallimento dal concetto di colpa, perché è vero che, soprattutto in periodi di crisi come questo, il fallimento o l'insolvenza non sempre derivano da una colpa dell'imprenditore, ma

La seconda è che si insiste sulla specializzazione del magistrato, che è fondamentale in questo tipo di processi, e si esplicita la necessità di un rafforzamento degli uffici giudiziari all'uopo preposti. È una cosa che diciamo spesso e il Ministro lo sa,

il Movimento 5 Stelle ha condiviso l'impianto generale e l'approccio del disegno di legge in esame, volto a riformare tutta la disciplina dei fallimenti e delle procedure concorsuali, condividendo la volontà di allontanarsi dallo stigma

alla necessità, secondo il nostro punto di vista, di conservare le competenze per le procedure concorsuali agli attuali tribunali ordinari. Sul punto avevamo

membri non togati, naturalmente aventi specifici requisiti di competenza tecnica, di esperienza e, soprattutto, di indipendenza, anche rispetto a situazioni di conflitto di interessi,

e che, per tali ragioni, possiedono comprovate capacità gestionali. Purtroppo questo nostro invito, rappresentato anche nell'ordine del giorno, non è stato compiutamente accolto dal Governo.

avrà un esito effettivo in norma, ma che per adesso è ancora fermo in Commissione - che prevede, come sappiamo, l'ampliamento della competenza delle sezioni specializzate dei tribunali delle imprese,

si prevede un aumento delle competenze del giudice onorario ed è facile immaginare che vi sarà un intasamento di molti tribunali circondariali cosiddetti medio-grandi, mentre quelli medi e piccoli finiranno per avere sostanziali cali nel contenzioso e nelle pendenze e c'è da temere che con la prossima non auspicata e denegata riforma della geografia giudiziaria, nella quale già si prevede che non necessariamente un capoluogo di Provincia debba essere sede di tribunale,

delle imprese e dei cittadini, che lamentano questo aspetto. La desertificazione giudiziaria, l'aumento dei costi dell'accesso alla giustizia civile ed amministrativa sono stati e sono, purtroppo, precisi obiettivi politici con cui questi Governi mirano a risolvere il problema dell'arretrato, del contenzioso e dei possibili procedimenti di infrazione avviati dall'Unione europea. Noi cerchiamo di contrastare questa politica legislativa

con la disposizione relativa ai tribunali, che rischia di scardinare in maniera definitiva l'equilibrio delicato dell'offerta e della domanda di giustizia sul territorio italiano e per questo motivo noi non potremo votare favorevolmente il disegno di legge

questo disegno di legge, che ha trovato anche la nostra collaborazione e il nostro appoggio, si basa su alcuni concetti fondamentali. In particolare, non solo noi sostituiamo il termine fallimento con il termine liquidazione giudiziale, giudiziale, ma vi è una attenzione particolare a quella che, signor Ministro, era una interpretazione forzata della magistratura negli anni Settanta quando, anziché dichiarare il fallimento rispetto alla crisi economica, risolveva la situazione con l'amministrazione controllata per avere, né più né meno, una possibilità di recupero della residua capacità lavorativa. Questa è la logica del disegno

Da un lato, è affermata la competenza territoriale, che è riferita al centro dei maggiori interessi del debitore. Dall'altro se si vuole veramente intervenire nelle situazioni che rappresentano anche possibilità di composizione della crisi dell'azienda, occorre non concentrare tutto nel tribunale delle imprese. Signor Ministro, la concentrazione nel tribunale delle imprese significherebbe, né più né meno, una deficienza di intervento giudiziario rispetto a quanto oggi viene assicurato. Per tale motivo io ho apprezzato, e come Gruppo di Forza Italia apprezziamo, la disponibilità espressa con il vostro parere favorevole al nostro ordine del giorno, ancorché con una riformulazione, che tiene conto della necessità

una distribuzione delle competenze capace di mantenere integra l'efficienza del tribunale delle imprese ma allo stesso tempo di garantire con la prossimità delle decisioni giudiziarie, che vi sia una partecipazione effettiva a quell'accertamento di possibili risoluzioni della crisi che occorre privilegiare. Io non dirò molto altro, perché gli emendamenti e gli ordini del giorno discussi questa mattina dimostrano che, quando vi è, indipendentemente dalla posizioni politiche di maggioranza e opposizione, la consapevolezza di operare nell'interesse del Paese, ci si adegua a determinate valutazioni confidando nella legittimità dell'impegno che il Governo ha assunto affinché si verifichino determinato situazioni.

Presidente, colleghi, signor Ministro, un'altra riforma arriva alla meta. Una riforma importante e strutturale; una meta attesa da anni: forse da troppi anni. Le procedure fallimentari, colleghi, erano legate a un altro mondo, sia economico che sociale che di assetto istituzionale. Eravamo legati alla legge fascista del regio decreto n. 267 del 1942,

Fallimenti e suicidi sono stati il tragico *leitmotiv* della crisi di questi anni. Come affrontare la crisi, anche dal punto di vista delle procedure concorsuali? Quale filo tenere in questo labirinto difficile e complesso? Ed ecco la riforma: una riforma che finalmente interviene in modo sistematico sulle procedure concorsuali finalmente in grado di confrontarsi con la brutta bestia della globalizzazione. La globalizzazione è in noi, demonizzarla non serve; subirla è sbagliato e ingiusto. La sfida aperta è governare la globalizzazione con regole moderne e capaci di fornire agli operatori economici un quadro armonizzato, almeno a livello europeo. Come il Ministro sa,

così come la chiusura di questa legislatura. Cari colleghi, il paradigma del fallito viene messo finalmente da parte:

attengono alla capacità dell'impresa di stare al passo con l'economia e le trasformazioni produttive. Ci dà anche un altro segnale importante e un altro insegnamento: l'impresa è un bene in sé. bene in sé. Ha un valore e si costruisce all'interno delle sue forze e delle sue qualità. L'impresa mette addirittura in discussione l'antico conflitto imprenditore‑lavoratore e immette all'interno delle sue dinamiche la capacità di cooperare e investire insieme, anche attraverso una condivisione delle responsabilità, dei profitti e delle perdite. Per queste ragioni la riforma è strutturale. Sposta l'asse delle procedure concorsuali sulla prevenzione, individuare il male prima che si concretizzi; occorre individuare le vie di uscita prima che producano un danno rilevante all'impresa e, quindi, all'imprenditore e ai livelli occupazionali. Bisogna accompagnare la crisi:

più magistrati specializzati e una migliore definizione delle competenze territoriali: una capacità, in sostanza, di presentare al nostro Paese

abbiamo dato importanza all'approvazione di questa strutturale e importante riforma. Ringrazio il relatore e tutti i Gruppi, perché in Commissione giustizia abbiamo lavorato insieme, e il Governo ha saputo recepire, attraverso gli ordini del giorno, alcuni punti che possono qualificare la legge in fase di approvazione delle deleghe. Ecco perché noi

Signor Presidente, volevo ringraziare il relatore, la Commissione e tutti coloro che sono intervenuti.

con un meccanismo distorto che ha macinato, nel corso di questi anni, molte risorse sia in termini di capacità imprenditoriali sia in termini di risorse legate ai beni materiali. Credo che con questo provvedimento si riesca non soltanto a rivedere, com'è stato detto, lo stigma, che spesso non è più giustificato in una economia globalizzata, ma a non sprecare neanche capacità imprenditoriale. Si può essere buoni imprenditori e avere avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice. un intervento positivo sull'utilizzo dei beni e sulle procedure, com'è stato ricordato. Vi è una focalizzazione su un punto che considero fondamentale: la ricerca della conservazione dell'attività d'impresa. Questo è un punto fondamentale per il nostro Paese. Noi ci allineiamo all'indicazione europea, ma lo facciamo tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema e dell'esigenza di costruire strumenti di autoanalisi per le imprese che, essendo spesso di carattere familiare, non sempre hanno quell'articolazione interna in grado di valutare le effettive condizioni finanziarie. Le procedure di allerta, per le quali, nell'esercizio della delega, avremo una particolare attenzione per tenere conto delle peculiarità del nostro sistema, consentono una autoanalisi rispetto all'andamento dell'attività imprenditoriale. Vorrei fare un'ultima considerazione: mi dispiace che non vi sia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle che si è

Non possiamo far sì che piccolissimi tribunali siano chiamati ad occuparsi di fallimenti che hanno dimensioni sproporzionate rispetto alla loro capacità di intervento reale e su questo punto non considero una desertificazione il fatto che si debbano fare magari 50 chilometri in più per rivolgersi ad una sede giudiziaria dove vi sia effettivamente una una specializzazione in grado di dare una risposta. Considero tutt'uno con la legge che stiamo approvando due provvedimenti che abbiamo già assunto e la legge ne consente un terzo: la partenza del registro dei crediti e dei debiti e il portale delle vendite. Per la prima volta in Italia abbiamo un portale unico di tutte le vendite che interessano i beni sottoposti a procedura di carattere fallimentare. È un passaggio fondamentale, perché significa avere dei prezzi omogenei nella valutazione dei beni, dopo anni nei quali lo stesso bene poteva essere valutato 5 in una Regione e 20 in un'altra Regione. Adesso abbiamo un ulteriore passaggio che sarebbe davvero il salto di qualità e che stiamo cercando di realizzare: costruire un mercato parallelo di tutti i beni sottoposti alle procedure fallimentari.

che credo sia nell'interesse delle imprese e del nostro Paese. Mi auguro che tutte le forze politiche raccolgano questo richiamo.

l'apertura di un dibattito a cui possono partecipare un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti, ovvero un'ora e quaranta

probabilmente in parte anche raggiunti e raggiungibili da parte del disegno di legge. Faccio cioè riferimento alla geografia giudiziaria e ai piccoli tribunali. Signor Ministro, lei ha fatto riferimento alla necessità che, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, i tribunali troppo piccoli potrebbero farsi carico di competenze e di procedure concorsuali, magari di particolare complessità o portata sociale, con un organico, competenze

come sempre accade quando si parla di argomenti tecnici e specifici, non solo dell'esperienza diretta di chi parla e di altri componenti del Gruppo, ma anche di *input* qualificati provenienti dall'esterno; in tal caso non ho difficoltà a fare riferimento all'organismo congressuale forense, che ha sollevato

venendo incontro alle possibili problematiche cui lei, Ministro, faceva riferimento, con un potenziamento di personale anche non togato, quindi anche non magistrati, in situazioni di massima trasparenza, di assenza di conflitto di interessi e di garanzia di professionalità e capacità; questa misura potrebbe verosimilmente far sì che il rischio che lei paventava possa non sussistere. A fronte di quest'impegno da parte del Governo, anche organizzativo e legislativo, ci sarebbe, sull'altro piatto della bilancia, la possibilità di dire alle nostre imprese, soprattutto a quelle piccole e in difficoltà,

istituzioni e del Governo. Ecco perché ho voluto approfittare del fatto che lei è entrato nel merito, dando soddisfazione ad alcuni punti, per avere la possibilità di rappresentarle quanto ho cercato di dire

Quel passaggio è importante. Ricordiamo che già attualmente, come si diceva prima, i tribunali delle imprese hanno avuto un aggravio e sicuramente un aumento delle pratiche attuali, dovuto anche al fatto che alcune modifiche normative hanno imposto che la procedura venga trattata davanti al tribunale delle imprese. Il dato preoccupante non è l'aumento delle pratiche e dei procedimenti in corso presso il tribunale delle imprese, ma i tempi per l'adozione delle decisioni, che

per rivedere l'impianto del codice civile. Ricordiamo che in quella riforma è previsto un grande aumento delle competenze dei tribunali delle imprese,

tenendo presente che il 25 per cento del totale delle giornate di lavoro perse è legato alla depressione. Era già dimostrato che l'assenza dal lavoro e il precariato sono associati a un maggior rischio di depressione. Su oltre 28 milioni di lavoratori, circa 6 milioni di italiani - uno su cinque - soffrono di *stress* da lavoro, con prevalenza delle donne. Oltre 3.200.000 sono le donne lavoratrici con problemi *stress*-collegati e disagi psichici. Di queste, circa un milione soffre di una condizione clinicamente rilevante e meritevole di un'attenzione specialistica, 500.000 per disturbi di ansia, 230.000 di insonnia e 220.000 di depressione. Tra i fattori determinanti vi sono le forti pressioni lavorative, le barriere culturali che rendono la carriera manageriale della donna più difficoltosa e impegnativa, ma soprattutto gli incarichi legati alla vita quotidiana e il ruolo di *care giver* all'interno della famiglia. La depressione è oggi la seconda malattia invalidante al mondo e si stima che nel 2030 sarà al primo posto, con altissimi costi sociali e un forte impatto economico. In base a tutto quello che ho affermato, ho apprezzato il disegno di legge Lorenzin, che prevede, tra le altre cose, che biologi e psicologi entrino a pieno titolo nelle professioni sanitarie. Vorrei che questo dettaglio non passasse inosservato e mi auguro che sia l'inizio di una piccola rivoluzione culturale attorno ad alcuni temi che mi sono estremamente cari. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento drammatico dei casi di depressione, oltre alla nascita di una serie di disturbi il cui minimo comune denominatore è quasi sempre lo *stress*. Il mondo di oggi ha evidentemente impostato dei ritmi che non per tutti e non sempre sono compatibili con una vita serena e con il ragionevole livello di benessere di cui ognuno ha bisogno per vivere. In questa era di velocità, relazioni superficiali, rabbia e guerre ideologiche è la mente a farne le spese, il nostro cervello, le nostre idee e i nostri sogni. Da un punto di vista clinico, questo può facilmente portare a un degrado delle condizioni psicofisiche che, se non viene individuato e curato in tempo, può assumere una quantità impressionante di forme, tutte negative. Il suicidio, estrema e tragica conseguenza di certi disturbi depressivi, è la parola che si tende a evitare, ma che indica un qualcosa che esiste e che è da combattere. Allo stesso modo, anche l'alimentazione come abitudine è andata sbiadendo, si è adattata ai ritmi imposti dalla società, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario. Un sano rapporto con il cibo è estremamente più possibile se anche questo si accompagna a una condizione psicologica serena. Quindi la depressione, in tutte le sue accezioni, è ancora oggi al centro di un dibattito culturale più che scientifico. Gli addetti ai lavori sanno perfettamente di cosa si tratta e conoscono la patologia e la gravità della situazione; tutti gli altri, però, spesso non la riconoscono come tale. Un soggetto depresso passa per una persona svogliata o che sta attraversando solo un periodo. di certe figure tra le professioni sanitarie è una presa di coscienza importante, a cui mi auguro possa seguirne una più sottile, ma anche più importante, sociale e culturale.